la Presidenza - nell'orario che sarà tempestivamente comunicato ai Gruppi - commemorerà la figura dell'ex senatrice Rina Gagliardi, recentemente scomparsa. Domani pomeriggio, in apertura di seduta, sarà commemorato Egidio Sterpa. Nel corso di questa settimana resta confermato l'esame del decreto-legge recante interventi urgenti in materia di energia e l'avvio dell'esame del disegno di legge di riforma universitaria. Per quest'ultimo provvedimento, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato differito alle ore 12 di domani. Si è inoltre proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Giovedì 22 luglio, alle ore 12,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. La chiama inizierà dai deputati. La seduta dell'Assemblea del Senato sarà sospesa intorno alle ore 14, per consentire ai senatori di recarsi alla Camera dei deputati, e riprenderà a conclusione della chiama dei senatori per il prosieguo dell'esame - anche con votazioni - degli argomenti all'ordine del giorno. Pertanto, lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo, già previsto per giovedì 22 alle ore 16, non avrà luogo. La prossima settimana, ore 16, non avrà luogo. La prossima settimana, i lavori dell'Assemblea riprenderanno martedì 27 luglio, alle ore 11,30, con il seguito dell'esame del disegno di legge di riforma universitaria. Nel corso della prossima settimana, che prevede sedute con votazioni fino al pomeriggio di giovedì 29 luglio e, se necessario, nella mattina dì venerdì 30, saranno inoltre discussi il decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, al momento all'esame della Camera dei deputati; il disegno dì legge in materia di sicurezza stradale, ove non riassegnato in sede deliberante; ratifiche di accordi internazionali, tra le quali la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori. In apertura della seduta pomeridiana di mercoledì 28 luglio, alle ore 16, si svolgerà la chiama dei senatori per la partecipazione al voto a scrutinio segreto mediante schede per 1'elezione di un componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciascun senatore riceverà una scheda nella quale indicare un solo nome. Dopo la chiama le urne resteranno aperte per consentire la più ampia partecipazione al voto. Tenuto conto della necessità di concludere i rilevanti argomenti previsti dal calendario dei lavori entro la sospensione per la pausa estiva, la Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente convenuto sull'esigenza che 1'Assemblea si riunisca nella prima settimana di agosto, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 2. Tra i provvedimenti che saranno calendarizzati alla ripresa dei lavori all'inizio del mese di settembre la Conferenza dei Capigruppo ha indicato il rendiconto e 1'assestamento del bilancio dello Stato, il bilancio interno del Senato e il disegno di legge collegato in materia di lavoro pubblico e privato.

Onorevoli colleghi, lo scorso 27 giugno è scomparsa prematuramente Rina Gagliardi, nostra collega nella passata legislatura. Nata a Pisa nel 1947, dopo essersi brillantemente laureata alla Normale, si trasferì giovanissima a Roma per sviluppare i suoi più grandi interessi: il giornalismo e l'attività politica. Nel 1971 aderì al gruppo de «il manifesto», che proprio in quell'anno si trasformava da rivista mensile in quotidiano, e si costituiva altresì come formazione politica, presentando una propria lista alle elezioni del 1972. Era l'inizio di una lunga carriera di redattrice della sezione politica de «il manifesto», del quale assunse anche, per un breve periodo, la direzione. Nella quotidiana attività di cronista Rina Gagliardi impegnava tutta la sua passione e la sua straordinaria capacità di analisi dei fenomeni politici, confrontandosi con acume e senso di apertura culturale anche con posizioni molto distanti dalla propria, e proponendo letture mai banali della realtà, come fu, ad esempio, per le sue riflessioni sugli effetti delle battaglie femministe nella politica e nella vita quotidiana. Dopo oltre 25 anni di collaborazione con «il manifesto», desiderosa di partecipare più direttamente alla contesa politica, passò prima a collaborare con il quotidiano "Liberazione", organo del Partito della Rifondazione Comunista diretto da Sandro Curzi, e successivamente accettò la candidatura al Senato nelle liste di quel partito nelle elezioni del 2006. Eletta quindi senatrice nella XV legislatura, fu componente della Commissione istruzione pubblica e beni culturali e della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico. La sua costante presenza ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e l'acume appassionato dei suoi interventi le guadagnarono in breve tempo la stima e la simpatia dei colleghi, rendendola nella considerazione generale una delle figure più autorevoli del Gruppo parlamentare e della sua parte politica. Oltre che ad offrire un prezioso contributo di pensiero e di passione ai più importanti dibattiti di quella complessa stagione parlamentare, il suo impegno quotidiano in quest'Assemblea fu rivolto in particolare alla difesa della cultura, e soprattutto - in coerenza con l'altra, grande passione della sua vita, accanto alla politica ed al giornalismo - alla tutela ed alla promozione della formazione musicale. La sua perdita priva il nostro Paese di una profonda intellettuale e di una lucida lettrice dei fenomeni politici e sociali, che non esitava a levare con coraggio, quando lo riteneva necessario, la sua voce critica verso amici ed avversari. Sono certo allora di esprimere i sentimenti di tutti i colleghi nell'invitare l'Assemblea ad osservare, nella memoria commossa di Rina Gagliardi, un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Signor Presidente, il ricordo della senatrice Gagliardi ci obbliga a ritornare a ritroso con il pensiero, perlomeno al forse addirittura prima, perché Rina Gagliardi fu una studentessa giovane e brillantissima che scriveva già benissimo quando era al liceo e che vinse un premio per il tema migliore sulla Resistenza prima ancora di terminare Poi frequentò la Normale, e lì dove manifestò la sua vocazione di lettrice e di studiosa critica. La sua vita è passata dentro l'esperienza de «il manifesto», un giornale scomodo, di lotta, di militanza sembra abbia scritto più di 2.500 articoli, il che denota, se ci si pensa solo un secondo, un'attenzione e una determinazione a cogliere nella sequenza del tempo - del quotidiano, della settimana, del mese la vicenda politica nel suo farsi con interesse, con "cattiveria", con capacità di penetrazione. Ma poiché il tempo stringe, penso che, se si deve raccogliere nel ricordo di un altro nome la sua la sua identità politica più intima, si debba qui ricordare quello di Rosa Luxemburg. L'attenzione che Rina Gagliardi dedicò a questa figura è anche emblematica del suo modo di intendere il comunismo: una lotta non necessariamente violenta (e tutti sappiamo che fine abbia fatto Rosa), una lotta determinata in nome dell'eguaglianza e dell'esercizio del pensiero critico, con una venatura pionieristica di femminismo, anche se forse per quella figura è ancora troppo presto per parlare di femminismo. Di fatto, con Rosa Luxemburg si realizza la costruzione, l'invenzione di una figura di donna come soggetto politico, al di là del sesso.

con capacità di studio e di sintesi, la figura di Rosa Luxemburg rende un po' la cifra specifica della sua attitudine politica e di studio: la passione per l'eguaglianza, la passione per i diritti, il il vietarsi la rinuncia alla lotta. La sua vita è passata attraverso un'antinomia precisa. Ha passato gli anni centrali nell'esercizio della libera critica, in un'esperienza come quella de "il manifesto" che non poteva essere che di disordine: il diritto di critica esercitato verso chiunque, verso tutti, verso tutte le idee, verso tutti i processi, verso tutti i partiti. Poi, ad un certo punto, c'è stato un momento di rapida transizione e di rottura: Rina Gagliardi è passata quasi di colpo dal ragionamento critico nel mondo del disordine -concedetemi questo termine - all'approdo alla quadratura di un partito, quasi come una sorta di rovesciamento del proprio atteggiamento precedente, quasi denotando la necessità di passare dal magma della confusione politica dei movimenti al bisogno di dare una quadratura alle cose. La scelta del Partito della Rifondazione Comunista arrivò come un punto di approdo di un cammino che ad un certo punto doveva esigere, per forza di cose, il concretarsi di un'idea di partito. Non potremo mai sapere se Rina Gagliardi si sia potuta ritenere soddisfatta di questo passaggio. Tuttavia, poiché la scelta della quadratura non è stata poi così felice e il cammino non è stato coronato da successi significativi, anzi, forse da una lenta dissoluzione, amo pensare che Rina Gagliardi, con la sua vocazione feroce e determinata nell'esercizio della critica, ad un certo punto forse avrebbe anche ripensato quest'altro passaggio come soluzione del suo tramonto, avrebbe preferito ritornare nel mare del disordine piuttosto che restare nell'ordine del partito, anche se mi rendo conto che questa è l'espressione di una

Signor Presidente, è con sincera vicinanza alla famiglia che, a nome del Gruppo della Lega Nord Padania, esprimo il più profondo cordoglio per la recente e prematura dipartita di Rina Gagliardi. vogliamo rendere omaggio ad una donna, ad una giornalista, ad una collega senatrice di indubbia raffinatezza intellettuale, una figura che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, lo scorso 27 giugno. Ricordiamo quindi Rina Gagliardi come una grande parlamentare una grande parlamentare che ha passato coerentemente la massima parte della sua vita nelle redazioni dei giornali di sinistra, a partire da «il manifesto», per passare poi a «Liberazione» e, fin dalla sua costituzione, alla testata «Gli Altri». Ci vorrebbero forse troppi aggettivi positivi - e non basterebbero - per provare a ricordare lo spessore umano e l'impegno professionale, oltre che ovviamente politico, della collega senatrice Gagliardi. A mio avviso il più significativo, proprio perché raro anche nel mondo della politica e delle aule istituzionali,

solo la coerenza può consentire ad una figura politica di essere al servizio delle istituzioni e non di mettere i ruoli istituzionali ricoperti al servizio della propria persona. Mi servirò dunque proprio di questo valore, di questo principio, del termine coerenza quale cordone ombelicale per ricordare le principali scelte che hanno caratterizzato la vita di Rina Gagliardi.

Fa parte del primo nucleo organizzato de «il manifesto» e coerentemente, nel 1971, quando viene fondato il quotidiano, si trasferisce a Roma per lavorare al giornale. Dal 2005 al 2006 diventa caporedattrice di «Liberazione», il quotidiano del Partito della Rifondazione Comunista, e con

Diviene quindi membro della 7a Commissione permanente istruzione pubblica, beni culturali di palazzo Madama, oltre a divenire componente della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico. In seguito allo scioglimento anticipato delle Camere e al disastro elettorale del 2008, lascia Rifondazione Comunista, ricominciando a tempo pieno e con la coerenza di sempre l'impegno giornalistico. Dal 2009, interrotti i rapporti con la testata di "Liberazione" collabora con diversi giornali, tra cui «Gli Altri», settimanale diretto da Piero Sansonetti. La sua mancata partecipazione all'istituzione parlamentare rappresenta ovviamente un addio alla politica istituzionale, che non ha però rappresentato, per nostra fortuna, un addio ai suoi coerenti contributi alla politica del Paese,

figura fondamentale quindi nel giornalismo e nel mondo della sinistra, anche e soprattutto per la sua cultura e la sua forte passione politica. Infine, la ricorderemo come una donna di intelligenza pungente e raffinata, sempre caratterizzata dal suo particolare intelletto e soprattutto dalla sua evidente coerenza. ricordiamo oggi Rina Gagliardi che per noi è stata collega ed amica. Io l'ho conosciuta giornalista parlamentare. In nessun modo perse le sue caratteristiche essenziali di curiosità, e può sembrare strano rispetto a quanti l'hanno dipinta come una donna dalle profonde, rigide convinzioni ideali, ma nessun passaggio, nessun tramutamento di Rina ci fu dal mestiere di giornalista a quello di parlamentare. Perché lei era, anche in ragione della sua straordinaria cultura, soprattutto una persona curiosa, profondamente curiosa. Io spiego così - e così se lo spiegano tutti coloro i quali l'hanno incontrata, l'hanno frequentata e le hanno voluto bene - il fatto che lei riuscisse ad intrattenere rapporti non formali con persone che erano distanti, e grandemente, dalla sua propria cultura politica e della sua stessa esperienza politica e di vita. Per Rina niente era mai stupido o banale, perché andava comunque a cercare il fondo delle cose, le ragioni per le quali alcune posizioni venivano assunte e, nella stessa attività giornalistica, l'incontro con un'altra persona non era, come qualche volta accade, l'incontro di chi già sa e deve farti dire ciò che tu hai pensato che pensi, ma era esattamente il contrario: un incontro vero, sincero, aperto, profondo e curioso delle ragioni per le quali quella persona avesse quell'idea o sostenesse quella posizione. In questo senso, prendeva davvero tutto molto sul serio, e ciò era sempre riconosciuto dall'interlocutore, nonostante il suo essere così evidentemente, solarmente ed orgogliosamente Non c'era nessun avversario politico (potremmo definirlo così in ragione del fatto che poi fu parlamentare

che agisse o chiedesse o si informasse o si incuriosisse in ragione di un pregiudizio, di un'idea che si era già fatta o di uno schema dal quale già partiva. In questo senso era, credo, la celebrazione di un modo di fare giornalismo e di interessarsi delle cose del mondo e della politica (che era il suo grande amore) talmente eccellente - adoperiamola, questa parola - da essere strano e raro ritrovarlo in altri soggetti. Lei sostanzialmente si divertiva: il suo modo di accostarsi al giornalismo e di fare la notista politica e il suo modo di fare il parlamentare era profondamente segnato dal fatto che ciò che faceva le piaceva moltissimo. E gli argomenti ai quali si appassionava vivevano di una passione vera, non di una simulazione di passione, mai di una simulazione di interesse. Altrimenti scattava l'ironia. È una cosa che mi ha sempre colpito di Rina: anche nei momenti più difficili, nei momenti dell'amarezza e della disillusione, non era mai né arrabbiata né remissiva, ma era la celebrazione del suo spirito arguto, cui l'amarezza diventava amara autoironia, divertente anche quella, come può esserlo esclusivamente l'autoironia delle persone davvero intelligenti e sincere nel non considerarsi il centro del mondo. Eppure era davvero molto più brava - molto più brava - di tanti altri. Abbiamo condiviso

in particolare di fronte alla bellezza della musica, da farne una persona davvero fascinosa. Il libro che lei ha scritto, «Devi augurarti che la strada sia lunga», ha un titolo che oggi in qualche modo ci intimorisce; alludeva certamente alla difficoltà, alla durezza

nell'affrontare una strada e un percorso che avrebbero potuto essere assai più lunghi del previsto. Il suo percorso è stato invece breve e si è chiuso in un lampo. A noi resta un grande rammarico, però credo che serva anche a noi giovarci, ancora una volta, della sua capacità di guardare

sono state dette delle cose talmente belle sulla senatrice e giornalista Rina Gagliardi che io mi limiterò ad forse quanto è stato detto; ma la sua personalità era così forte e preponderante che tutti l'hanno colta da tutti i punti di vista. Rina Gagliardi è stata una voce storica ed autorevole della sinistra italiana. Ha seduto nei banchi di quest'Aula, è stata eletta senatrice senatrice di Rifondazione Comunista nel 2006, ma prima di tutto è stata una grande giornalista: una giornalista dal carattere tenace, dall'intelligenza puntigliosa e pungente, stimata dai compagni, ma molto anche dagli avversari politici. Il giornalismo è stato per lei una delle forme della politica: si fa politica sedendo in quest'Aula, si fa politica anche - e in modo molto incisivo - facendo del giornalismo. I giornalisti che seguono i lavori parlamentari la ricordano spiritosa e anche molto sarcastica, come tutti i toscani, ma soprattutto una fonte preziosa non solo di notizie, ma di interpretazioni ed analisi delle situazioni politiche. Nella sua vita ha fatto un'infinità di cose. Da giovane sessantottina comunista, più che da Marx, Lenin e Gramsci, è stata affascinata da Rosa Luxemburg, alla quale ha dedicato la sua tesi di laurea appena laureata nella mitica "Normale" di Pisa, ha lasciato la sua città per venire a Roma ed entrare poco più che ventenne a «il manifesto». Inizia così nei primi anni '70 una storia che dura quasi trent'anni, fino al 1997 quando, con profonda amarezza, rompe il rapporto con il quotidiano del quale nel 1986 è stata direttrice insieme a Mauro Paissan. Rileggere gli oltre 2000 suoi articoli dice Valentino Parlato - è come leggere una storia del nostro Paese, dagli scontri sociali e politici, alle roventi polemiche culturali. Rina Gagliardi è un'intellettuale e una donna coltissima, che ha letto tutto e ricorda tutto, grazie anche a una memoria che si può definire prodigiosa.

La sua non è solo una curiosità intellettuale, ma anche umana - come è già stato detto - nei confronti di chiunque incontri: politici, metalmeccanici, femministe, studenti, sportivi. Cultura e passione sono - secondo Massimo D'Alema - i tratti dominanti della sua personalità. C'è passione nello strappo, nella rottura, con «il manifesto». Passione per la sua irrinunciabile indipendenza intellettuale, per la libertà di pensare che la determinano a scrivere, nell'ottobre 1997: «Dissento profondamente dalla posizione assunta da "il manifesto" sulla crisi del Governo Prodi». Motivo dello scontro è la caduta del Governo provocata dal voto contrario di Rifondazione Comunista: «il manifesto» si è dichiarato per la conservazione del Governo Prodi, il che per Rina Gagliardi, che rifiuta di cedere a compromessi, segna - sono sue parole "la separazione del giornale dalla sua anima radicale". Successivamente, su "Liberazione", che dirige con Sandro Curzi, scrive editoriali molto importanti, spesso controcorrente. Ultimamente collabora alla testata «Gli Altri», diretta da Piero Sansonetti, e a «Il Riformista» di Antonio Polito. Ma nella vita di Gagliardi, oltre al giornalismo, alla cultura, alla politica, vi sono altre due passioni: innanzi tutto quella per la musica, sia essa classica, sinfonica, lirica o pop;

anticonformista, rimasta prima di tutto per tutta la vita sempre fedele a sé stessa, sono certa che gli amici, i compagni, i colleghi politici e gli avversari, conserveranno l'immagine forte, indimenticabile e viva di quanti l'hanno conosciuta. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare ha comunicato che, nella seduta del 20 luglio 2010, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la circoscrizione Estero - ripartizione Europa: Raffaele Fantetti e Claudio Micheloni. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

il provvedimento in esame reca una serie di norme transitorie dirette ad assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole nel periodo di intenso traffico estivo, nelle more del completamento delle procedure di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione Spa e della Come è noto, il 3 novembre 2009 un accordo tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate ha permesso il passaggio del controllo delle società regionali marittime da Tirrenia alle Regioni di riferimento: Caremar alla Campania, Saremar alla Sardegna e Toremar alla Toscana. Il processo di privatizzazione di Tirrenia e della controllata Siremar, società che assicura i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, avviato da Fintecna, è in fase di avanzata realizzazione. lo stato di incertezza che condiziona il buon esito della procedura ha determinato, nelle ultime settimane, difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e Siremar, e una situazione in cui gli amministratori della società hanno ritenuto di non utilizzare anche alcune linee di credito già in essere. La principale finalità del decreto consiste, allora, nel garantire la situazione finanziaria di Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione Pertanto, l'articolo 1, lettera *a)*, del provvedimento, derogando allo statuto di Tirrenia e Siremar, nonché alle pertinenti norme del codice civile, rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro cinque giorni

Si prevede poi, alla lettera *b),* che la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti ed i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica, dagli amministratori unici e dagli altri organi di amministrazione e controllo di Tirrenia e di Siremar resti a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti viene esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei suddetti soggetti, dei dipendenti pubblici e dei soggetti titolari di incarichi pubblici. La lettera *c)* stabilisce che fino al 30 settembre 2010 o, se anteriore, fino al perfezionamento della privatizzazione, le banche e di altri intermediari autorizzati possano erogare a Tirrenia nuovi finanziamenti, così come la quota non ancora erogata di finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942. in caso di successive procedure concorsuali che dovessero attivarsi qualora la privatizzazione di Tirrenia non sortisse esito positivo, le banche e gli altri soggetti finanziatori sarebbero pagati prima di tutti gli altri creditori, compresi quelli privilegiati. I creditori suddetti non hanno diritto di voto in sede di eventuali procedure concorsuali e sono esclusi dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo e dalla percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Gli atti, le garanzie ed i pagamenti relativi ai nuovi finanziamenti non sono soggetti ad azione revocatoria. Si impone a Tirrenia il vincolo di utilizzare i nuovi finanziamenti esclusivamente per far fronte ai bisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente ovvero per finanziare, per le stesse finalità, la Siremar Spa. Infine, la lettera *d)* stabilisce che la garanzia prestata da Fintecna per le linee di credito derivanti dai nuovi finanziamenti sia subordinata alle condizioni e ai termini previsti dalla normativa comunitaria recata dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009. La garanzia prestata da Fintecna si rende necessaria per assicurare i finanziamenti che, ordinariamente, le società Tirrenia e Siremar riescono a reperire sul mercato e che invece, nella situazione transitoria che precede la privatizzazione, non sono più assicurati dalle banche. L'articolo 2 del provvedimento individua nel giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* la data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, quest'ultimo è in vigore dallo scorso 8 luglio e - come poc'anzi evidenziato - sono già decorsi i cinque giorni ed è già avvenuta la nomina dell'amministratore straordinario. minoranza*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la relazione del collega Musso, quale si è attenuto con grande competenza alla lettera del decreto. Credo tuttavia che l'occasione odierna ci obblighi a parlare del processo più generale di privatizzazione della Tirrenia,

che ha come azionista di riferimento un ente pubblico; credo che non vi siano precedenti nella storia europea di un simile modo di aprirsi al mercato e alla concorrenza. Sarebbe anche interessante capire cosa pensa Bruxelles di questo percorso di privatizzazione. Inoltre, ritengo importante fare, sia pure brevemente, un po' di storia ed un po' di ordine nella vicenda. Oggi funziona più o lo Stato copre con sovvenzioni di equilibrio (un eufemismo molto elegante) quanto la Tirrenia e le consorelle perdono annualmente, cioè tutto il *deficit* di cassa viene coperto

numerosi competitori in questo ambito. In realtà, l'Unione europea non chiedeva *tout court* di privatizzare; eccepiva, invece, sul sistema della convenzione considerata un aiuto di Stato. Facciamo un po' di chiarezza anche sul sistema delle convenzioni.

per il servizio universale e per la continuità territoriale con le isole. In realtà, i conti del vice ministro Vegas sono - per così dire - un po' a spanne. Sono andato a spulciare con maggiore precisione i conti ed ho verificato un dato decisamente più preoccupante: nel 2007, a fronte di 292 milioni di euro di ricavi, la Tirrenia ha avuto 46 milioni di euro di sovvenzioni; nel 2008 i ricavi sono diminuiti a 279 milioni

Le società regionali, di cui si parlava prima (toscana, campana e così via), stanno anche peggio: nel 2007, a fronte di ricavi complessivamente di 81 milioni di euro, hanno ottenuto sovvenzioni per 135 milioni

nuovo indirizzo per il servizio pubblico doveva essere avviato ed in questo senso c'è un forte intervento dell'*Antitrust* che, con riferimento alla Regione Campania - ma in realtà è un monito che può essere esteso all'insieme del servizio di trasporto su mare - chiede una più chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico e una messa a gara dell'assegnazione dei sussidi; e questo è anche il monito dell'Unione europea. In questo quadro si situa il percorso indicato di privatizzazione: privatizzazione: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo, il decreto-legge n. 135 del 2009 e finalmente, il 22 dicembre, l'invito di Fintecna a manifestazioni

è l'unica società regionale che, pur data in dono alla Regione Sicilia, la Regione ha rifiutato di acquisire, cosa importante da tener tener presente per un giudizio complessivo su questa vicenda); un pacchetto di sovvenzioni particolarmente lucroso, perché per Tirrenia si prevedono 73 milioni annui di sovvenzioni per un totale di 584 milioni per gli otto anni e per Siremar di 56 milioni, per un totale di 672 milioni per i 12 anni. Si tratta, in totale, di un miliardo e 256 milioni di aiuti pubblici per chi si aggiudicherà l'asta per la privatizzazione di Tirrenia. Certo, nell'indicazione c'è anche la garanzia per il servizio pubblico, per la continuità territoriale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

a questo debito c'è anche un piccolo patrimonio, in particolare una bella collezione d'arte di Tirrenia, da Savinio a Sironi, a Fiume, a Pomodoro e ad altri artisti italiani; ma non è l'arte che attrae gli investitori, anzi l'unico investitore: è evidente che l'unico interesse dell'operazione è l'accaparramento del flusso miliardario di sovvenzioni pubbliche. Questo è il vero bottino a disposizione.

può stare in piedi una società con questo squilibrio patrimoniale? Nel mondo normale, credo di no. Siamo dunque di fronte ad un evidente *flop* annunciato, un disastro, quello della Tirrenia, che non sembra trovare una soluzione, anzi è facile prevedere che i guai per i passeggeri si aggraveranno. C'è poi un forte tam tam di queste ultime ore, signor Presidente, colleghi del Governo e della maggioranza: se

siamo di fronte a un "piano B" come diceva il vice ministro Vegas? Si va verso lo spezzatino in tante gare diverse per le varie rotte oppure no? È facile quindi prevedere un'estate di fuoco. È evidente che il Governo ha operato in questo percorso con grande leggerezza e con grande approssimazione, ha portato la nave di Tirrenia tra Scilla e Cariddi con un rischio di naufragio che è evidentemente molto alto: un bel capolavoro! apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, nel dichiarare aperta la discussione generale, avverto che da parte del Governo è stato presentato l'emendamento 1.0.100 in materia di autotrasporto.

la norma che era stata approvata in Commissione bilancio in sede di esame della manovra finanziaria e che poi fu espunta

è assolutamente evidente - e certamente non le sfuggirà, signor Presidente - che il testo stesso è improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento. È evidente che la materia recata daell'emendamento stesso, che riguarda la disciplina dell'autotrasporto per conto terzi su gomma (una vera e propria riforma, o controriforma: riforma, o controriforma: a seconda dei punti di vista) non ha nulla a che vedere con il contenuto proprio di questo decreto che riguarda, al di là dell'indicazione testuale del contenuto del decreto recata dal titolo, esclusivamente Tirrenia, o meglio la gestione transitoria di Tirrenia nelle more della privatizzazione. Che cosa c'entri l'autotrasporto con Tirrenia è un mistero che vorremmo ci Infatti, signor Presidente, lei ebbe ad adottare un orientamento per noi assolutamente soddisfacente (se non ricordo male, il 20 novembre del 2008) in materia di ammissibilità degli emendamenti, in particolare in sede di conversione

quei principi che la Corte Costituzionale ha così chiaramente enunciato verrebbero totalmente svuotati di contenuto. anche di un ulteriore e delicato profilo, che lei conosce molto meglio di me, signor Presidente, ossia che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione in legge dei decreti-legge non va fatta solo in relazione al contenuto proprio del decreto, ma anche rispetto alla valutazione dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge. Ci troviamo di fronte ad un caso assolutamente particolare, poiché il Governo ‑ come ci è noto ‑ ha già deliberato un decreto-legge su questa materia, che è all'esame della Presidenza della Repubblica. Quindi, oggi il Governo intende seguire una via che è assolutamente irrituale e per noi inaccettabile. La preghiamo, signor Presidente, di pronunciarsi nel senso dell'improponibilità di questo emendamento, dichiarando sin d'ora la nostra assoluta disponibilità ad un esame celere di questo provvedimento, che pure ha la sua importanza. Sappiamo che a monte vi è un accordo tra le categorie professionali noi può discutere, ma noi siamo disponibili a consentire un vaglio rapido di questo provvedimento nella Commissione di merito, sia che si decida di proseguire sulla via della emanazione del decreto-legge, sia che si voglia presentare un disegno di legge, magari anche discutendolo in sede deliberante. Perché no! Saremmo disponibili a valutare anche questa opportunità, per garantire un ordinato svolgimento del procedimento legislativo.

attinenti a materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pari del decreto-legge all'ordine del giorno, concernente anch'esso la regolarità dei trasporti, seppur marittimi. Pertanto, questa Presidenza ritiene l'emendamento proponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per le ragioni già illustrate questa mattina ai Capigruppo, che ne hanno preso atto quando l'emendamento è stato preannunciato, con l'intesa che i Gruppi avrebbero avuto un congruo termine per la presentazione di subemendamenti, termine fissato per le ore 20 di questa sera. Il decreto-legge, al di là della Tirrenia, parla di trasporto, seppur marittimo, ma il tema affrontato è quello del trasporto; quest'emendamento affronta il tema del trasporto ed ecco perché questa Presidenza lo ritiene ammissibile. Non possiamo in alcun modo accettare la sua decisione

Ripeto, signor Presidente. Lo stesso obiettivo che il Governo vuole conseguire con questo provvedimento lo si conseguirà ancor più se il provvedimento stesso seguirà la via scelta dal Governo, che è quella del decreto-legge, che non siamo noi a chiedere, Consiglio dei ministri ha deliberato qualche giorno fa: il Governo ha deliberato un decreto-legge identico a questo testo, sottoponendolo all'esame del Presidente della Repubblica. Oggi, in un provvedimento che non riguarda affatto la materia, infila questa norma nei modi ai quali stiamo assistendo. Ciò è inaccettabile, signor Presidente. È un precedente, o meglio, una decisione che contraddice la sua interpretazione, che corrisponde alla nostra, del Regolamento. È una violazione

La storia è abbastanza nota, Presidente. *(Brusìo).* Mi chiedo se lei voglia che io legga l'intera relazione che abbiamo già condiviso con i membri della Giunta

Grazie Signor Presidente, la vicenda riguardante il senatore Guzzanti è relativa ad un articolo che egli ha scritto su un quotidiano a tiratura nazionale, denominato "Il Giornale", il 31 ottobre 2003, a valle di una sentenza di un tribunale italiano che si riferiva a uno dei processi interessanti il senatore presidente Giulio Andreotti. A seguito di questo articolo, venne sporta querela dal dottor Caselli, il quale, nell'ambito di un procedimento penale dinanzi al tribunale di Monza, si oppose, alla sua difesa, alla richiesta della difesa del Guzzanti di vedere eccepito l'articolo 68 della Costituzione. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato il fascicolo processuale, ha ascoltato il senatore Guzzanti e ha potuto verificare che gli argomenti contenuti all'interno dell'articolo che «il Giornale» pubblicò il 31 ottobre 2003 si riferivano a materie più e più volte affrontate dall'allora senatore Guzzanti. Abbiamo indicato, all'interno della relazione, numerosi atti di natura strettamente parlamentare, che il senatore Guzzanti ha redatto personalmente o che ha sottoscritto o che ha concorso a redigere. Quindi, alla Giunta è sembrato di poter proporre all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni dell'onorevole Guzzanti, Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Vi è solo da aggiungere, per concludere, signor Presidente, che tale deliberazione è stata assunta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità

dichiaro di non condividere le conclusioni della Giunta testè illustrate dal collega Lusi. il senatore Guzzanti definisce il processo Pecorelli, in cui rimase coinvolto il senatore Andreotti, un'invenzione, una costruzione del

poiché il dottor Caselli non era certamente in servizio presso la procura della Repubblica di Perugia ma, evidentemente, presso quella di Palermo, attribuirgli

ha provveduto a querelare il senatore Guzzanti. Senza entrare nel merito, è evidente che quanto costruito

Presidente, come Popolo della Libertà, senza voler andare per le lunghe, anche perché la relazione è stata abbondantemente supportata e suffragata da elementi obiettivi, condividiamo le conclusioni del relatore.

Signor Presidente, molto telegraficamente, mi rimetto alla relazione e alle conclusioni che sono state rassegnate, anche perché concordate dalla Giunta. Su queste conclusioni si è registrata la convergenza della Giunta e quindi sostanzialmente ritengo non vi siano altri elementi da aggiungere.

parlamentari è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento in cui è parte l'onorevole Mantovano, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione Chiedo al relatore, senatore Lusi, se intende intervenire.

è legata ad un procedimento civile, più esattamente ad un atto di citazione che un candidato consigliere comunale alle elezioni del 2008 ha depositato presso il tribunale civile di Roma, chiamando come convenuto il senatore Mantovano in relazione ad alcune affermazioni che lo stesso avrebbe fatto, scritto e inviato attraverso un'agenzia di stampa, ma che, a detta dell'attore, non risulterebbero corrispondenti alla realtà dei fatti. Da un approfondito esame che è seguito all'audizione del deputato Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, oggi onorevole Sottosegretario, e dall'acquisizione del fascicolo processuale in sede civile abbiamo potuto verificare non solo un discordanza enorme tra le dichiarazioni rese dall'attore in sede di atto di citazione e la documentazione a riscontro della stessa, ma anche alcune profonde differenze tra i fatti che assurgevano a fondamento dell'accusa - ancorché, ripeto, stiamo parlando di un procedimento civile nei confronti del deputato Mantovano, senatore all'epoca dei fatti - e quanto effettivamente avvenuto. veniva dichiarato dall'attore che il senatore Mantovano lo avrebbe accusato di non aver sottoscritto un documento, mentre poi si è riscontrato che nell'atto di citazione l'attore stesso parlava di un documento che è stato sottoscritto quattro anni prima, con un altro Ministro, in una condizione in cui i fatti non coincidevano assolutamente. Volendo astrarci dalla verifica fattuale, poiché teoricamente non comporterebbe alla Giunta di entrare nel merito di questa vicenda, ci ha interessato verificare se le attività del senatore Mantovano all'epoca dei fatti si erano occupate di immigrazione di extracomunitari e di tutte le questioni per le quali l'attore lo accusa nell'atto di citazione. La Giunta, avendo potuto verificare che vi sono ben 11 atti

costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli,

limitare semplicemente a dei brevissimi cenni esplicativi dovendo, tra l'altro, rappresentare all'Aula un ulteriore elemento sopravvenuto, sia pure irrilevante ai fini della deliberazione che compete al Parlamento. è facilmente deducibile dalla relazione, il 14 maggio 2010 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli

n. 361 (concorso in scambio elettorale); 110, 61, n. 2, del codice penale, 223, primo e secondo comma, n. 2, seconda ipotesi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta);

La Giunta ha poi concluso, a maggioranza, per il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. sindacato che compete al Parlamento è relativo *in primis* all'accertamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa il cosiddetto *fumus persecutionis* nell'ambito del procedimento nel quale si agisce nei confronti del parlamentare; in subordine, dove si dovesse ritenere

All'esito degli approfondimenti istruttori svolti, ed audito anche il senatore Nespoli, la Giunta, sia pure a maggioranza, ha concluso nel senso citato, ravvisando più che un ragionevole dubbio circa l'esistenza del *fumus* e, in ogni caso, ritenendo che non ricorrano le circostanze di assoluta eccezionalità per cui, laddove per ipotesi - e così secondo la Giunta, ancorché a maggioranza, non è questo ragionevole dubbio non sussistesse, comunque sarebbe consentita l'applicazione della misura. In telegrafica sintesi e rimandando alla relazione, credo che sia doveroso illustrare all'Aula l'ambito della vicenda nella quale si procede. Trattasi di vicenda di carattere concorsuale, quindi di natura fallimentare, che si colloca anni prima rispetto al momento in cui si comincia ad indagare nei confronti del senatore Nespoli,

corso di un colloquio che si svolge e viene intercettato ambientalmente nello studio del curatore fallimentare ad anni di distanza dal fallimento medesimo.

del proprietario effettivo della società. Questa chiamata in correità è di fatto il filo conduttore di tutto il percorso accusatorio nei confronti del senatore Nespoli. giusto quindi che l'Aula del Senato sappia che questa chiamata in correità - che poi si articola nella serie di ipotesi accusatorie contenute nel provvedimento che, anche per quanto riguarda l'esplicitazione dei singoli capi di imputazione, è a disposizione di tutti per rapidità di esposizione mi richiamo - non ha trovato alcun oggettivo riscontro; anzi, semmai c'è da dire che, se ci sono stati riscontri, sono stati di segno contrario. Vi è poi un altro elemento che ha indotto la Giunta a riflettere adeguatamente sul perché si volesse prima chiedere e poi disporre una misura cautelare in ordine ad una vicenda datata anni prima, che vede buona parte della sua dimensione di carattere bancario, finanziario ed economico palesemente ricostruibile *per tabulas* - perché evidentemente così è - e al tempo stesso con un'oggettiva serie di

di fatto impossibile. Basterebbe pensare a questo presunto scambio elettorale che, per quanto riguarda il senatore Nespoli, sarebbe stato assolutamente privo di alcuna motivazione, posto che altro era il suo collegio nel 2001 e che nel 2006, com'è noto, il sistema elettorale non determinava alcuna di queste possibili cointeressenze in sede di scambio elettorale. Quindi, la Giunta si è posta il problema di comprendere come mai, di fronte ad un quadro siffatto, ovverosia chiamata in correità assolutamente e palesemente interessata, che si colloca ad anni di distanza dall'inizio di una vicenda concorsuale ampiamente documentabile non suffragata di alcun riscontro, anzi significativamente smentita in alcuni passaggi, basata tutt'al più su dei «sentito dire», di fronte ad alcune accuse che di per sé erano prive di logica e verosimiglianza - sarebbe sufficiente illustrare da questo punto di vista all'Aula (altro aspetto) il presunto sviamento di clientela in relazione ad una società che si occupava di vigilanza privata e che, avendo perso per la mancata contribuzione previdenziale, il decreto prefettizio era di fatto inoperante e privo di valore

volendo anche superare quello che per la maggioranza della Giunta rappresentava sicuramente il primo invalicabile limite a concedere l'autorizzazione della misura, si poneva il fatto che non vi era né pericolo di fuga, né di inquinamento di prove, tenuto conto di tutto ciò che vi ho detto, né di reiterazione di condotte, atteso che si tratta di fatti legati ad una società fallita anni prima. Detto tutto ciò, e sia pure nei limiti del sindacato che ci compete, e proprio perché costituisce, ad avviso del relatore, utilissimo elemento di riscontro per comprendere come quel dubbio fosse ragionevole, va segnalato che lo scorso 6 luglio, cioè in epoca successiva all'espressione della Giunta e alla successiva redazione della relazione,

all'Aula: il GUP del tribunale di Napoli, su richiesta dello stesso pubblico ministero Piscitelli procedente, ha assolto colui che secondo l'impalcatura accusatoria, quella del chiamante in correità l'amministratore di questa società, era l'uomo del quale si serviva il senatore Nespoli all'interno della società, essenziale e necessario in ordine agli stessi reati. Solo in questi limiti, che sono quelli di di riscontrare come a valle di ciò che la Giunta aveva già in qualche modo individuato come motivo di più che ragionevole dubbio, si colloca un fatto che, almeno ad avviso sommesso del relatore, è *tranchant* sul punto, ripeto, il 6 luglio, su richiesta dello stesso pubblico ministero, il GUP di Napoli, in un procedimento connesso a carico di chi, secondo il chiamante in correità, era essenziale al senatore Nespoli per la commissione dei reati che gli vengono contestati - e quindi, se non li ha commessi lui, a maggior ragione non può averli commessi il senatore Nespoli - quest'ultimo è stato assolto per non avere commesso il fatto. Il pubblico ministero, ad avviso del relatore, avrebbe dovuto necessariamente chiedere la revoca della misura cautelare. Non averlo fatto, in questo contesto ed essendo lo stesso pubblico ministero procedente, determina più che un ragionevole e fondato dubbio circa l'esistenza di un *fumus persecutionis*.

Signor Presidente, fatta riserva di una richiesta specifica in ordine a quest'ultima segnalazione del relatore Mugnai, il mio intervento sarà essenzialmente di carattere giuridico. Vorrei ricordare innanzitutto come nella Costituzione repubblicana, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'immunità parlamentare non si configura come un diritto soggettivo del singolo parlamentare, ma come una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità, che può concederla o meno sulla base di una sua valutazione politica. Tradizionalmente, la valutazione politica dell'Assemblea (e della Giunta proponente) è stata ricollegata all'esistenza di un *fumus persecutionis* che giustificava il diniego di autorizzazione a procedere, quando tale istituto era vigente (prima del 1993). In proposito, si era più volte sottolineata la marginalità applicativa di un criterio interpretativo che considerasse il *fumus persecutionis* in termini strettamente soggettivi, riconducibili cioè all'esistenza di un *animus persecutionis* da parte del magistrato procedente. Fu per questo motivo che, sempre sotto la vigenza del precedente istituto autorizzatorio, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella seduta del 16 giugno 1988, approvò un documento nel quale si dichiarava che «con l'espressione s'intende (...) persecutoria l'azione penale che, per il tempo e le modalità del suo esercizio ovvero per la sua manifesta infondatezza, pur diretta nei confronti del singolo parlamentare, costituisca un *vulnus* per l'istituzione parlamentare». La schematizzazione che ne derivava nella pratica delle Giunte induceva a distinguere tra: *fumus persecutionis* di primo grado, ovvero la persecuzione dolosa del magistrato nei confronti del parlamentare; *fumus persecutionis* di secondo grado o soggettivo, quando deriva dalle modalità e dal tempo dell'esercizio dell'azione penale; *fumus persecutionis* di terzo grado o oggettivo, che emerge dalla manifesta infondatezza dell'azione. Abolita l'autorizzazione a procedere, un effetto di trascinamento interpretativo ha indotto a ritenere che i medesimi criteri potessero essere trasposti all'azione cautelare penale, nell'ambito della quale sono inoltrate alle Camere di competenza le richieste di autorizzazione cosiddette *ad acta*, per provvedimenti coercitivi nei confronti dei parlamentari. Non è ininfluente considerare l'effetto pratico che questa trasposizione aveva nel procedimento penale. È ben vero che era sempre puntualmente ribadito, nella relazione della Giunta di diniego dell'autorizzazione alla misura cautelare, che «Certamente la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione procedimentale della sussistenza o meno delle esigenze cautelari tipizzate dall'articolo 274 del codice di procedura penale; né per converso la Giunta deve automaticamente far discendere un *fumus persecutionis* da un accertamento incidentale della mancanza di tali esigenze cautelari». Aggiungo: anche per non consentire pratiche difensive anomale o abnormi quali quella di utilizzare e strumentalizzare in sede processuale la valutazione della Giunta e del Senato in materia di *fumus persecutionis*. Per correggere allora quella deformazione, che rischiava tra l'altro di attribuire un vantaggio improprio all'inquisito, alterando la serenità degli organi giudicanti sul merito degli addebiti, non è bastato innalzare il livello dell'accertamento operato dal Parlamento in termini di probabilità e di possibile strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare. È stato invece necessario ripensare il criterio con cui la Giunta stessa operava ispirando la considerazione che assolutamente non interferissero con il procedimento pendente. Questo per così dire nuovo criterio è stato definito alla Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura, dopo una disamina dei numerosi casi (oltre cinquanta) di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature. Tale nuovo criterio è stato confermato sia nella XIV che nell'attuale legislatura. Il criterio da seguire è stato ed è tuttora quello di un bilanciamento tra gli elementi indicati dai magistrati nell'ordinanza cautelare, come il grave indizio di colpevolezza per reati di particolare gravità e la dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari, e l'esigenza l'esigenza che, salvo casi eccezionali, la Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alla Costituzione. In materia di misure restrittive della libertà personale, un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato vuole che l'integrità dell'organo parlamentare costituisca il fine prevalente della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68 della Costituzione, che può essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, sono tali da soverchiare l'altra esigenza. E in tal senso si sono pronunciati sia la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo che la Corte costituzionale, anche molto di recente. Ricordo che quando la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, allora presieduta da Giorgio Napolitano, esaminò la *ratio* dell'istituto immunitario esistente nei Paesi membri, affermò che "nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi ed immunità, il Parlamento" - ovviamente nazionale - "mira principalmente a sostenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e a garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni". la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 188 del 2010, è intervenuta nello stesso senso nella seguente maniera, recitando: «E' opportuno, innanzitutto, considerare che l'avere il legislatore costituzionale (articolo 68 della

in luogo dell'originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento - individuato soltanto alcune specie di atti del procedimento penale per compiere i quali verso un parlamentare è prevista l'autorizzazione della Camera di appartenenza (cosiddetta autorizzazione *ad acta*), rende palese che non già e non più l'intero procedimento, ma solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare, e che queste sono suscettibili di sacrificio nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di

spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare... e per converso - la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta...che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta,

oggi ci viene proposta stravolge questo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, riprendendo il vecchio concetto di *fumus persecutionis* e, leggendo la relazione del senatore Mugnai, ci rendiamo conto di tutta una serie di contraddizioni perché, se da una parte dice che non spetta alla Giunta sostituirsi al giudice, però, subito dopo, effettua un'ampia esposizione che lo porta a dire che esiste un dubbio sulla sussistenza del *fumus persecutionis.* E qui addirittura introduce un concetto giuridico nuovo: quello del *fumus* del *fumus* Inoltre, il relatore non parla mai del criterio di necessità, così come ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza parlamentare. Invece, ciò che va contestato è proprio questa mancata esposizione nei termini dovuti del criterio di necessità che impone alla Camera di negare l'autorizzazione *ad acta* solo qualora il bilanciamento, in concreto, tra esigenze di salvaguardia della funzione parlamentare, da un lato e, dall'altro, funzione di accertamento dei reati, di tutela delle vittime, di obbligatorietà dell'azione penale e di garanzia della sicurezza dei cittadini, propenda inequivocabilmente in favore delle prime. In questo senso, c'è anche una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (si vedano i casi Cordova, De Jorio, Cofferati). Nell'effettuare questo bilanciamento, peraltro, il Parlamento non può appropriarsi di funzioni rimesse esclusivamente all'autorità giudiziaria. La relazione avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali intende disattendere la valutazione fornita dalla magistratura circa la necessità dell'autorizzazione all'arresto, non limitandosi ad invocare questo generico *fumus* del *fumus persecutionis*, non supportato da alcun elemento di fatto. Ciò che avrebbe dovuto fare la relazione sarebbe stato, in conclusione, valutare se effettivamente l'interesse all'integrità della composizione dell'Assemblea parlamentare potesse, nel caso specifico, essere legittimamente sacrificato a fronte di un'imputazione per reati gravissimi, quali la bancarotta fraudolenta aggravata ed il riciclaggio, considerando altresì che impropria sarebbe una pretesa di limitare l'autorizzazione solo alle prove cui sia attribuibile il carattere della decisività, al cui concetto non può essere ridotto e circoscritto quello di necessità. Parole queste con le quali la Consulta, con la sentenza del 2010 ricordata, ha ribadito come le Camere non possano negare l'autorizzazione *ad acta* solo in ragione della presunta non decisività della prova, in quanto la valutazione in ordine all'esigenza di disporre un determinato atto di indagine (sia esso una prova, sia esso una misura cautelare) non spetta al Parlamento, ma all'autorità giudiziaria. In conclusione, non sono assolutamente condivisibili le osservazioni e la conclusione cui perviene il relatore di maggioranza, motivo per cui non potremo che votare contro la proposta da lui formulata.

puntuali che il collega Casson ha enucleato con grande attenzione, è evidente che il *fumus persecutionis* nel caso in specie non vi è e non è rintracciabile in alcunché. E d'altra parte, anche il relatore altro non ha fatto se non arrampicarsi sugli specchi per giustificare l'esistenza del *fumus persecutionis*. Egli infatti ha cercato - e lo ha fatto - di entrare nel merito del procedimento che interessa il senatore Nespoli, tentando di puntualizzare una serie di fatti ed episodi che non interessano nell'Aula parlamentare: noi dobbiamo soltanto mettere in evidenza che non vi è, da parte dei magistrati del tribunale di Napoli, alcuna volontà

un gruppo di senatori del Partito Democratico, a nome del proprio Gruppo, avendo effettuato un'istruttoria accurata in Giunta delle immunità, propone, in difformità dalle conclusioni del relatore, di dichiarare la insussistenza del cosiddetto *fumus persecutionis*. cercare di spiegare che l'indagine a carico del senatore Nespoli non riguarda soltanto lo stesso senatore Nespoli, ma un numero più vasto di persone, le quali in sono già state destinatarie di provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale. un'indagine ampia, che riguarda il voto di scambio, la bancarotta, fatti che hanno cagionato il fallimento di un'importante società di vigilanza campana, campana, la distrazione di fondi, la falsificazione di quietanze bancarie a danno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (mi fa piacere che oggi sia qui presente anche il Ministro del lavoro che, sotto questo profilo, potrebbe costituirsi parte civile nel provvedimento) ed il riciclaggio di somme abbastanza ingenti. Per sostenere che vi è un intento persecutorio, bisognerebbe innanzi tutto dimostrare che nelle indagini tempi, modalità ed azioni dei

del senatore Nespoli e che raccontano - noi non giuriamo sulla verità di questo racconto - di un sistema di commistione tra affari, politica e strumentalizzazione di organizzazioni

non è per il voto di scambio che viene chiesta la misura cautelare a favore del senatore Nespoli: il pubblico ministero lo esclude, proprio perché si tratterebbe di fatti risalenti molto indietro nel tempo.

In tutto questo, nella sequenza degli atti e nella sequenza temporale delle indagini, non vi è nulla che faccia pensare ad un accanimento giudiziario nei confronti del nostro collega Nespoli.

proponendo alla Giunta di deliberare sul fatto, per noi dirimente, che non si tratta di un'indagine montata. Poi può darsi che l'indagine non arrivi a nulla; può darsi che un giudice terzo, domani o dopo, dica che non ci sono le condizioni per condannare, bensì per assolvere, ma intanto il Parlamento esca dalla facile strada del processo al processo. La teorica del *fumus persecutionis* non è altro che questo: cercare di fare, senza contraddittorio tra le parti (nella Giunta delle immunità, come sapete, si leggono carte e si ascolta il senatore),

ascoltare e valutare l'esigenza del Senato di garantirsi la sua piena operatività, che però è una valutazione successiva a quella sul *fumus persecutionis*

con la ricostruzione che il senatore Mugnai ha fatto dell'intera vicenda rassegnandola a questa Camera. Camera. La seconda parte delle sue argomentazioni, quelle che riguardano appunto l'applicazione del cosiddetto criterio del *plenum* del Senato, avremmo voluto discuterla in Giunta, avremmo voluto discuterla in Giunta, sulla base del tipo di autorizzazione a misura cautelare richiesta, dei possibili tempi d'esecuzione della misura, del ruolo del senatore Nespoli in Senato; avremmo voluto anche ragionare in maniera innovativa

coperto da questo duplice timbro: *fumus persecutionis* che cancella tutto e poi alcune argomentazioni, in parte condivisibili, sul mantenimento del *plenum* del Senato. Se invece sarà approvato l'ordine del giorno proposto all'Aula dal Gruppo del Partito Democratico, Partito Democratico, si dice che non c'è *fumus persecutionis* e si rimandano le carte alla Giunta per decidere sull'applicazione in concreto dei criteri di salvaguardia della prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

brevemente, anche perché il relatore, senatore Mugnai ha, con la sua consueta chiarezza espositiva, illustrato all'Assemblea la relazione, con tutti gli argomenti,

alcuni aspetti che confermano la sussistenza del *fumus persecutionis*, elemento del quale bisogna necessariamente tener conto secondo una corretta interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione del regime di garanzie che la norma costituzionale introduce a tutela del Parlamento. In questa vicenda, come illustrato dal relatore e come emerge dagli atti, vi sono sicuramente elementi sintomatici del *fumus persecutionis*, a cominciare dalla circostanza che, ad esempio, il pubblico ministero non ha trasmesso tutti gli atti relativi alle indagini espletate, non consentendo quindi al giudice che ha poi formalizzato la richiesta del provvedimento di avere conoscenza del quadro completo. In tal senso, ad esempio, manca la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dall'ispettore di polizia, la dottoressa Coppola, a proposito della necessità che gli istituti di vigilanza siano assoggettati alla disposizione sulla tenuta del cosiddetto registro degli affari, circostanza, questa, che nell'impianto accusatorio complessivo ha assunto una particolare rilevanza. Un'altra anomalia è quella relativa all'attribuzione ad un dipendente, tale Esposito di Castellammare di Stabia, della circostanza che alcuni dei posti dell'istituto di vigilanza sarebbero stati assegnati come strumento di pressione o di favore verso taluni richiedenti, ma dalle indagini è emerso che nessuno, tra le centinaia dei dipendenti dell'istituto, aveva questo cognome, e soprattutto che nessun dipendente con questo cognome proveniva da Castellammare di Stabia. Quindi, la fonte accusatoria indicata come essenziale è poi risultata, all'esito delle indagini, inesistente. Come pure manca il riscontro a proposito delle dazioni che sono state riferite, ma non provate, e le stesse operazioni finanziarie tra società riferibili al senatore Nespoli o a familiari del senatore Nespoli rispetto all'istituto di vigilanza La Gazzella si è poi verificato, dalla stessa consulenza disposta dal pubblico ministero, essere unidirezionali, nel senso che questi movimenti sono stati in direzione dalle società all'istituto e non viceversa. viceversa. Infine, a proposito delle indagini espletate, è emerso che le stesse trattative per la cessione dei contratti, che sono state poi indicate a proposito del danno economico, patrimoniale che sarebbe stato arrecato all'istituto, in realtà, sono state avviate e concluse solo dopo la revoca dell'autorizzazione prefettizia; quindi, quando l'istituto aveva cessato ogni attività e comunque non era più abilitato a condurre alcuna attività. La cessione dei contratti ha posto al riparo l'amministrazione residuale dell'istituto da azioni di risarcimento che i titolari dei contratti avrebbero potuto agevolmente espletare per la mancata esecuzione del servizio. Quindi, abbiamo un quadro di figure sintomatiche, a proposito del *fumus* *persecutionis*, elemento importante che, unitamente

concorre sicuramente a corroborare le conclusioni della relazione relativamente al diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza. Gruppo del Popolo della Libertà, esprimiamo convintamente voto favorevole alle conclusioni rassegnate dal relatore della Giunta.

ricordo che, poiché la Giunta propone il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare, coloro che sono favorevoli al diniego coloro che sono favorevoli al diniego voteranno sì, premendo il tasto verde; coloro che invece sono favorevoli alla concessione dell'autorizzazione voteranno no, premendo il tasto rosso;

premendo il tasto bianco. In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

con ricorso del 16 dicembre 2009, il tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 1534/08 RG, pendente

confermo le conclusioni della Giunta essendo la probabilità di vincere il ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale praticamente nulla e anche in forza dell'invito perentorio che viene dal Governo agli organi costituzionali di questo Paese di risparmiare danari a favore dell'abbattimento del debito pubblico e di utilizzazioni più utili. Per tali ragioni, riteniamo che si possa, prima, ma si debba evitare la costituzione del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione: oltre che per il risparmio, anche per evitare una brutta figura, stante la consolidata giurisprudenza della Corte in merito a fattispecie

anche perché in effetti dobbiamo ricordarci la originaria deliberazione di insindacabilità adottata sempre dalla Giunta nella seduta del 19 febbraio. Quindi, l'interesse a resistere nel conflitto di attribuzione, che ha per oggetto appunto la delibera di insindacabilità medesima, che ha adottato l'Assemblea del Senato, ha necessità di essere confermato. Non mi tratterrei più a lungo su questo argomento, ma ritengo che assolutamente il Senato debba assumere una deliberazione di costituzione in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e per il tramite anche di un avvocato del libero foro, perché

della strada che si è immaginato di intraprendere, che era quella di affidarci all'Avvocatura dello Stato. Affido questa mia riflessione, che per la verità abbiamo già affidato alla sua forte e antica sensibilità, presidente Schifani, di verificare ulteriormente se fosse praticabile quella strada, ma del fatto che il Senato debba costituirsi in giudizio, non già per tradizione o per antico retaggio, ma per ottemperare al deliberato già del 19 febbraio del 2009, ne sono assolutamente convinto. Quindi, noi senatori del Popolo della Libertà riteniamo di dover

le conclusioni della Giunta che si è espressa a maggioranza in senso contrario alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio.

La Giunta ha concluso nel senso di non doversi il Senato costituire in questo giudizio; il senatore Sanna ha insistito sulle conclusioni della Giunta; il senatore Izzo ha dichiarato, invece, di non condividere tali conclusioni. Passiamo

con la quale quell'Assemblea ha ritenuto di poter qualificare i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli, deputato e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, oggetto di procedimento penale pendente presso il tribunale ricorrente, come riferibili all'articolo 96 della Costituzione e ha quindi negato l'autorizzazione a procedere all'autorità giudiziaria. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 giugno 2010, depositata in cancelleria il successivo 11 giugno e notificata al Senato il 30 giugno 2010. Nella seduta del 13 luglio 2010, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto. La Giunta ha, inoltre, manifestato il proprio avviso favorevole a che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge dell'11 marzo del

il ministero e senza l'intervento, né dell'Avvocatura dello Stato (che, come sappiamo, resiste a prestare a favore delle Camere questo tipo di servigio) né dei professionisti del libero foro, cioè degli avvocati. Abbiamo notato che, nelle nostre costituzioni, come in quelle della Camera, la rappresentazione delle ragioni del Parlamento molto spesso segue, quasi parola per parola, le pregevoli relazioni che la Giunta o l'Assemblea del Senato, con l'ausilio dei competenti uffici del Senato della Repubblica, propongono alla nostra discussione e alla nostra deliberazione. Noi proponiamo, quindi, che in termini adesivi al ricorso sollevato dalla Camera (la Camera si costituisce, ovviamente), il Senato aderisca sì al ricorso ma in in forma diretta, utilizzando il privilegio, che il legislatore di oltre 50 anni fa ha dato agli organi dello Stato, di potersi costituire direttamente; e che il Senato devolva, come

Non cambia nulla in termini di qualità di intervento del Senato, perché noi abbiamo dei documenti che rappresentano l'eccellenza nella prospettazione delle tesi del Parlamento e, intanto, inviamo un segnale al Paese di credibilità della politica e anche - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - di adesione ad un sistema che imporrà agli organi costituzionali, negli anni a venire, un risparmio netto del 10 per cento rispetto ai loro costi. Iniziamo da qui.

Presidente, vorrei molto brevemente soffermarmi sulle conclusioni in merito alla scelta della costituzione in giudizio in questo conflitto di attribuzione, cui, dopo un approfondito dibattito, è pervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Innanzitutto, la Giunta ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di prendere parte al giudizio, e questo anche in ragione delle complesse questioni giuridiche che sono sottese alla vicenda, correlate anche ad un'altra questione sulla quale l'Assemblea già si è pronunciata esattamente un anno fa, in occasione dell'esame della posizione del senatore Castelli. Su quella vicenda è intervenuta la stessa Corte costituzionale con un'importante sentenza e quindi questo giudizio, e l'intervento adesivo che il Senato si accinge a dispiegare in questo contenzioso, appare oltremodo opportuno. Personalmente, ma anche a nome del mio Gruppo, nutro delle perplessità sull'ipotesi della costituzione in giudizio senza avvalersi dell'assistenza di uno o più avvocati del libero foro. Non sfuggono le ragioni dell'interpretazione del combinato disposto degli articoli 20 e 37 della legge sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, che il senatore Sanna ha prima ricordato e più diffusamente illustrato nel corso della discussione in Giunta, e che hanno trovato accoglimento nelle conclusioni della stessa. Vorrei però a questo punto dare lettura proprio dell'ultimo comma dell'articolo 37 della legge citata, che dispone: «Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiono personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori». In sostanza, la legge offre un'alternativa a ciascuno degli organi dello Stato che hanno diritto ad intervenire in giudizio, cioè o quella di farsi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori oppure quella di comparire «personalmente». Tuttavia, non è un caso che sino ad oggi, ed in maniera concorde, le Assemblee legislative in sede di conflitto abbiano sempre optato per la prima ipotesi, dunque facendo ricorso a rappresentanti del libero foro, questo per una serie di ragioni che sinteticamente proverò a ricordare, in quanto molti sono i dubbi connessi all'interpretazione della facoltà di comparire personalmente che la norma riconosce a taluni organi dello Stato. In primo luogo, non è chiaro, ed in particolar modo non lo è per il Senato, anche in relazione alle norme del suo Regolamento e soprattutto in ragione della sua funzione di organo legislativo, se la possibilità di comparire personalmente implichi anche la possibilità di scegliere e di individuare qualsiasi soggetto, ad esempio anche un senatore, che rappresenti in giudizio l'organo costituzionale. In secondo luogo, andrebbe poi accuratamente valutata la praticabilità di comparire per il tramite degli Uffici del Senato. Poiché, infatti, si può dubitare che quest'ultima sia da intendersi come una comparizione "personale", proprio perché parliamo degli uffici, si dovrebbe verificare se non sia necessario disporre, nell'ambito degli uffici e dei soggetti che negli stessi vengono poi designati alla rappresentanza, di avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, come del resto dispone l'articolo 20 della legge sul funzionamento della Corte costituzionale. Pur senza addentrarmi nel merito della valutazione cui è pervenuta la Giunta, penso però che il Senato non sia ora nella condizione di approfondire adeguatamente il tema, che è gravido di una serie di valutazioni e di implicazioni anche sulla stessa ritualità e regolarità dell'eventuale costituzione in giudizio prodotta in questo modo. È un'ipotesi interessante, sulla quale si potrà tornare con più tempo e con maggiore calma per condurre gli approfondimenti necessari. Ora però la perentorietà del termine per la costituzione in giudizio induce quest'Assemblea a seguire la via ordinaria, quella che è stata sempre praticata e che in passato è stata anche pacificamente e concordemente seguita dalla Camera dei deputati, oltre che dal Senato della Repubblica. In base, quindi, a queste considerazioni, avanzo la proposta di una soluzione difforme dalla seconda parte delle conclusioni rassegnate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità In definitiva, se l'Assemblea deciderà per la costituzione in giudizio del Senato, propongo che questo sia rappresentato, come di consueto, da uno o più avvocati del libero foro. Circa, infine, l'esortazione che il senatore Sanna ha ripetuto questa sera qui in Aula - ma che era argomento già trattato nel corso dei lavori della Giunta - al contenimento delle spese, esistono molti altri rimedi, che sono stati anche in quel dibattito ricordati, come la possibilità che al momento del conferimento dell'incarico vi sia la sottoscrizione di convenzione con una mitigazione, per così dire, del tariffario professionale. Tutto ciò, naturalmente, è rimesso al prudente apprezzamento della Presidenza che saprà, con la consueta saggezza, assumere anche in questa vicenda la soluzione e la scelta più opportuna per tutelare il superiore interesse del Senato. Grazie a lei,

Se tale proposta risulterà respinta, la Presidenza sarà autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero foro.

Colleghi, potete stare seduti? Mi state dando le spalle. Per favore, vi potete sedere? Non chiudo la votazione sin quando i senatori non sono seduti.

banchi del Governo. Vedo soltanto il ministro Bondi che ha votato ed è presente

a Stava, in Trentino, crollavano gli argini di un doppio bacino di raccolta dei fanghi prodotti dalla lavorazione della fluorite e nella vicina miniera della Montecatini. Una marea di fango e di detriti percorse tutta la Val di Stava per quattro chilometri, fino alla confluenza con la Val di Fiemme e con il fiume Avisio. Furono travolti alberghi, abitazioni, segherie, malghe, case coloniche. Persero la vita 268 persone fra valligiani, turisti, lavoratori di diverse Regioni italiane impegnati sia nella miniera, sia negli alberghi e nelle altre località turistiche. Fu una sciagura annunciata, signora Presidente, o peggio prevista, a causa dell'incredibile precarietà degli argini in terra battuta che contenevano le migliaia e migliaia di tonnellate di residui fangosi e melmosi della miniera, ma a causa anche della mancanza totale di manutenzione da parte della società Montecatini. Dopo 25 anni le famiglie delle vittime oggi si dichiarano soddisfatte per quanto riguarda il risarcimento materiale, ma chiaramente altrettanto non possono dire per quanto riguarda la perdita morale dei propri cari. L'angoscia di allora per interi nuclei familiari inghiottiti dal fango è l'angoscia di oggi. Come responsabili di quel disastro finirono sotto processo dieci persone: furono condannate da due a cinque anni di reclusione, ma, come accade spesso in Italia, nessuna di loro affrontò un solo giorno di detenzione. Alle cerimonie commemorative che si sono svolte fra sabato e ieri hanno partecipato anche delegazioni del Vajont - quindi di Longarone - e di Cavalese, a memoria delle due sciagure del Cermis, la funivia che cadde per due volte, anche in questo caso per colpa dell'uomo. In conclusione, si tratta di un percorso della memoria purtroppo ricco in Italia, bisogna fare in modo che il dolore, che rappresenta la memoria costante e la compagnia quotidiana della gente che abita in quelle vallate, appartenga un po' a tutta la comunità nazionale. Questo è l'appello che mi è stato affidato in questi giorni, cioè di fare in modo che l'Italia non dimentichi una sciagura della portata di quella di Stava: per questo ho chiesto di portarne la memoria in quest'Aula e

finestra"). Riguardano la situazione del carcere di Marassi: una situazione assolutamente drammatica, da molto tempo drammatica. Pensate, nelle condizioni attuali e con il caldo che c'è,